Comunico che in data 5 luglio 2024 è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il seguente disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia: «Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia (1183)», già presentato alla Camera dei deputati il 4 luglio 2024.

Signor Presidente, colleghi e colleghe, la 10a Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 1161 di conversione del decreto-legge n. 73 lo scorso 12 giugno e ha svolto un fitto ciclo di audizioni con l'intento di procedere ad un esame accurato del testo da concludere nei tempi previsti. Attualmente la Commissione è impegnata nella fase della trattazione degli emendamenti ed è stata convocata anche nella giornata di ieri con la previsione di lavorare ad oltranza proprio allo scopo di portare in Aula oggi il provvedimento. Come è noto, il decreto-legge contiene norme di grande delicatezza, su alcune delle quali è aperta la dialettica con le associazioni di categoria

La necessità di giungere ad una delicata composizione degli interessi, che presumibilmente sfocerà nella stesura di talune norme interamente sostitutive di quelle oggi presenti nel provvedimento d'urgenza, unitamente a ragioni di correttezza e al rispetto istituzionale, non hanno dunque né consigliato né permesso di concludere l'esame in Commissione in tempo utile per la seduta dell'Assemblea di stamattina, il cui ordine del giorno, Presidente, come lei sa, è stato stilato ed elaborato oltre dieci giorni fa. Nell'attesa degli esiti del richiamato confronto, mi riservo dunque di modulare di conseguenza i lavori della Commissione da me presieduta, la quale potrà presumibilmente consentire al relatore di riferire all'Aula nella giornata di domani.

Non ce l'ha perché il Governo non è in grado in questo momento di trovare risposte a un'esigenza fondamentale, ossia quella di garantire ai cittadini un accesso rapido e sicuro alle cure di cui hanno bisogno. che sia fondamentale oggi rendersi conto che questa incapacità del Governo si ribalta totalmente sulla qualità della vita delle persone. Non penso che si possa risolvere il tema delle liste d'attesa soltanto con un decreto e credo che ciascuno di noi, come forza politica, sia chiamato a un atto di responsabilità propria, perché tutti abbiamo governato, tutti sappiamo quanto sia difficile risolvere i problemi della sanità e tutti dobbiamo concorrere a trovare le soluzioni giuste per risolvere una volta per tutte il tema delle liste d'attesa. Certamente però questo balletto sui provvedimenti, a cui ci sta ormai abituando il Governo per questioni esclusivamente politiche e di rotture all'interno della maggioranza che ci governa, credo che sia inaccettabile. È inaccettabile che in Commissione

vogliamo richiamarlo con forza. Ringrazio il presidente Zaffini per i tentativi che sta facendo in Commissione, però credo che anche il Parlamento, sia da questa che dall'altra parte, dovrebbe dare un segnale al Governo. Non si può continuare a fare decreti *spot*, che non risolvono i problemi,

Signora Presidente, noi denunciamo - e mi fa piacere che sia presente il ministro Ciriani - la totale mancanza di attenzione da parte del Governo sui lavori del Parlamento. Come il ministro Ciriani sa, la settimana di lavoro delle Commissioni era stata prevista per consentire l'esame del numero in questo momento spropositato

in alcuni casi inutili, tant'è vero che alcuni di essi saranno assorbiti da altri (e non lo abbiamo deciso noi, come è noto, ma lo ha deciso la maggioranza, rinnegando sé stessa). Questo numero sproporzionato di decreti aveva inevitabilmente portato ad attività - lo dico al presidente Malan e al presidente Romeo - che di fatto finivano in un imbuto, in una Commissione più che in altre, perché stava lavorando su un decreto molto delicato, il cosiddetto decreto-legge sulle liste d'attesa, stante la grandissima condizione di sofferenza in cui si trova la sanità pubblica italiana. Bene, la scorsa settimana, presidente Zaffini, lei ha sconvocato tutte le sedute della Commissione. Non è stato possibile, per la 10a Commissione, fare un'ora di dibattito nel merito degli emendamenti, per l'assenza del Governo. Noi abbiamo contestato questa condizione e abbiamo chiesto -

si comunicano all'inizio dei lavori della Commissione, non aspettando l'esito dei pareri del Governo, perché non siamo al mercato, presidente Zaffini, ministro Ciriani, siamo a Palazzo Madama. Abbiate rispetto per l'opposizione. Se noi presentiamo le nostre tesi, abbiamo la necessità di sapere se il Governo non le condivide, se ci sono dei problemi procedurali e se

Questa commissione, per la quale siamo tutti condizionati da chissà quali motivi, noi non l'accettiamo. Presidente Zaffini, le dico che lei non è un autocrate, ma un Presidente di Commissione; lei non può dire - Presidente, mi rivolgo a lei perché poi

Tra l'altro, non sto toccando l'articolo 2, che è l'oggetto vero della discussione; sembra quasi che la maggioranza non voglia discutere dell'articolo 2. Su questo poi apriremo una discussione seria in Commissione; lo stanno facendo le nostre colleghe, ma lo faremo certamente ancora in Aula. Ebbene, la relazione illustrativa - non scritta dal Partito Democratico, signora Presidente, ma dal Servizio bilancio - afferma che «per il rifinanziamento negli anni successivi» - sto parlando del potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche specialistiche - «si farà riferimento alle relative leggi di bilancio annuali». Il Servizio bilancio sottolinea che la copertura degli oneri delle leggi dovrebbe essere approntata in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, non potendosi rinviare le coperture alle successive leggi di bilancio. Questo dovrebbe - lo dico al Presidente della Commissione bilancio, che non vedo - avere almeno il parere della 5a Commissione; lo dico ai colleghi della 5a Commissione: dai miei modesti ricordi e in base

ad una settimana dal voto, per rispondere chiaramente al no detto a Montecitorio *(Applausi)* al disegno di legge Schlein che dava un'indicazione di rotta. Potete non condividerla, ma non potete dirci che non possiamo nemmeno presentare gli emendamenti, perché questa è la condizione in cui siamo, con la maggioranza che ci dice: questo è l'emendamento del PD, non lo guardo nemmeno. Questa cosa è inaccettabile e non è scritta in nessuna parte del Regolamento. Chiudo, signor Presidente, con la sottolineatura di un ossimoro che è sotto gli occhi di tutti: l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, l'assunzione di personale per il ricorso alle prestazioni aggiuntive, lo svolgimento di attività sanitaria in orario notturno, prefestivo e festivo, gli indispensabili adeguamenti tecnologici e gli aggiornamenti informatici, necessitano di un'adeguata disponibilità di risorse economiche e di personale. Questo è ciò che evidenzia la Conferenza delle Regioni e delle Province nel parere negativo espresso su questo decreto-legge l'11 luglio Presidente Romeo, non è cambiato nulla. Io non so cosa sta accadendo in queste ore nella Conferenza Stato-Regioni e se si è aperto un improbabile suk dentro la maggioranza, ma una cosa posso garantirle: le Regioni nella loro interezza e la Conferenza all'unanimità, se il Governo non torna indietro dopo queste valutazioni, non potranno che essere unite contro una forzatura che è sotto gli occhi di tutti e che contestiamo. Quindi, mi auguro, signor Presidente, che domani mattina i colleghi della 10a Commissione, dopo aver lavorato e dopo essersi confrontati, possano mettere l'Aula nella condizione di fare una discussione seria che il Paese aspetta da ventuno mesi.

i decreti cadono sugli scogli della realtà: è quello che sta accadendo in questi minuti. Se torniamo indietro di qualche settimana con la memoria, questo decreto-legge è stato presentato dal Governo in piena settimana elettorale, con toni trionfalistici, con i quali si annunciava agli italiani che, grazie a questo provvedimento, si sarebbero finalmente risolte tutte le problematiche attorno ad una vicenda gravissima, gravissima, come quella delle liste d'attesa, che ha messo in discussione il diritto alla salute dei nostri cittadini. Dopo un mese, la maggioranza viene in Aula e dice che non ha ancora creato le condizioni per convertire questo straordinario provvedimento che avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi dei nostri cittadini. Nella sua retorica molto circospetta e diplomatica, il presidente Zaffini ci ha detto che è in corso una dialettica, che - tradotto in maniera forse un po' più comprensibile - significa che stanno litigando, signora Presidente. Stanno litigando furiosamente all'interno della maggioranza e non ci voleva la zingara per capire l'interpretazione data dal ministro Schillaci. A proposito, dov'è dov'è il ministro Schillaci, dov'è il sottosegretario Gemmato? Noi abbiamo visto che in Commissione non si sono presentati non sono venuti in Parlamento. Lasciano il ministro Ciriani, come una sorta di neo-cireneo, costretto a dover portare un peso che non è naturalmente addebitabile alla sua personale personale o istituzionale responsabilità. Insomma, il ministro Schillaci, in maniera stentorea e tipica di una parte della maggioranza, aveva inserito all'articolo 2

ma le ASL. Se la singola ASL della Provincia più lontana dell'impero non avesse rispettato le prerogative stabilite sulla base del rispetto dei parametri per le liste d'attesa, ecco che il prode Schillaci sarebbe intervenuto in forza di legge con un proprio decreto, e avrebbe esercitato la sua azione risolutiva, non si capisce bene come, visto che non sono state previste risorse e visto che questo tema era palesemente incostituzionale, per risolvere il problema della ASL della Provincia dell'impero. Dopodiché che cosa è accaduto? C'è stata la sommossa di tutti i Presidenti delle Regioni, perché perché mentre voi ci state spiegando che c'è l'autonomia differenziata per tutti, vi siete dimenticati che esiste una Costituzione vigente che stabilisce che queste competenze sono delle Regioni, e poi, naturalmente, abbiamo visto che una forza di maggioranza, la Lega, con il suo Capogruppo, ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 2, cioè del cuore di questo decreto. Siccome state ancora litigando, non siete in condizione di venire in Aula per dirci come proseguire. Ma da quello che si evince sembrerebbe che la soluzione mediana sia in qualche misura riferibile alla sceneggiatura che Pietro Germi e Monicelli fecero di uno straordinario pezzo cinematografico degli anni Settanta e Ottanta del nostro Paese. Mi riferisco naturalmente alla figura del conte Mascetti, che io qui non ripeterò. Tuttavia ci venite a dire che la soluzione di tutto questo è la creazione di nuova burocrazia, con un acronimo terribile, il responsabile unico dell'assistenza sanitaria

perché non avete competenze, perché non avete soldi, perché non avete idee. Questo è il motivo vero per il quale non stiamo andando avanti. *(Applausi)*. Se questo decreto-legge avesse davvero avuto necessità e urgenza, noi l'avremmo convertito nella settimana della campagna elettorale, perché se veramente avesse avuto la capacità di poter intervenire, con i soldi oltre che con le organizzazioni reali,

veniamo a sapere da altri livelli. Vorrei dire in quest'Aula, signora Presidente, che tutti hanno avuto in mano la griglia degli emendamenti, tranne i parlamentari competenti: le sembra normale che in questo Paese noi dobbiamo venire a sapere da terzi

però in questi casi le incongruenze e i pasticci politici ogni tanto vanno in collisione, quindi noi stiamo bloccati per una questione meramente politica

il Governo si sente in qualche modo messo in discussione. Ma allora perché facciamo le audizioni? Perché ascoltiamo i pareri delle persone più competenti di noi? Questo è quello che sta avvenendo

lo abbiamo già detto e ripetuto e lo ripeto un'altra volta - si arriverà alla mortificazione dell'attività parlamentare e quindi del ruolo che il parlamentare deve avere nella costruzione delle proposte di legge, mantenendo distinto chi è all'opposizione e chi è al Governo. Questo, però, è un dato che tutti siamo chiamati a rispettare.

del decreto, ma vorrei ricordare che il tema delle liste d'attesa non è solo - visto che sono stato tirato in ballo come firmatario di un emendamento - rappresentato dal decreto che è in discussione. Arriverà anche il disegno di legge, quindi l'intervento in di due provvedimenti e questi ritardi sono semplicemente dettati dal fatto che il Governo, proprio a seguito della bocciatura

che tenga conto dell'obiettivo che il Governo si è prefissato con i controlli sul tema delle liste d'attesa, naturalmente rispettando il principio di autonomia delle Regioni. Questo è quello che sta succedendo.

qual è il prodotto, il frutto di questo dialogo, e dopo si esprimeranno eventualmente i vari giudizi politici. L'emendamento della Lega non aveva l'obiettivo di colpire, come è stato detto da qualcuno, il cuore del provvedimento. Aveva solo l'obiettivo di favorire il dialogo tra il Governo e le Regioni. Ve l'abbiamo spiegato in tanti

colleghi, io volevo solo brevemente rispondere ai colleghi riguardo a dei passaggi procedurali in Commissione. Nel merito del provvedimento,

al comma 3 così recita: «Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente»: inappellabilmente. E al comma 1, sempre l'articolo 97 recita che: «Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti». A questo riguardo, la differenza con il Regolamento dell'altro ramo del Parlamento probabilmente induce qualche volta a qualche valutazione poco pertinente. Riguardo all'assenza del Ministro, attraverso il suo tramite, tramite, signor Presidente, mi rivolgo al collega Borghi per ricordare che il Ministro è venuto nell'aula della Commissione personalmente a illustrare il decreto, all'inizio della discussione.

Già nel 2019, «Il Sole 24 Ore» diceva che le liti tra Stato e Regioni impegnano una sentenza su due della Consulta. Questo, ovviamente, a causa della modifica del Titolo V, che è stata fatta un po'

Signor Presidente, mi pare che il presidente Zaffini abbia spiegato in modo esaustivo tutte le questioni che sono state sollevate. mi sembra che l'operato del presidente Zaffini sia sempre stato ineccepibile, portando avanti i lavori su provvedimenti molto importanti, come questo,

si trovano di fronte alle difficoltà delle liste d'attesa. Le modalità del cammino parlamentare di questo provvedimento sono state illustrate dal presidente Zaffini e il ritardo è principalmente dovuto all'interlocuzione, che è sia per lealtà istituzionale, sia per approfondire quali competenze siano delle Regioni e quali invece dello Stato. Credo dunque che siamo in una situazione di normalità tutto sommato ritengo anche normale che le opposizioni attacchino su questi punti e stigmatizzino i ritardi. Tuttavia, non c'è nulla che non abbiamo già ampiamente visto: ritardi nell'arrivo dei pareri, ritardi nell'andamento e nell'inizio dell'esame in Assemblea, cose che abbiamo già visto in molte legislature, forse in tutte.

indubbiamente genera problemi che toccano in modo molto importante le vite di tante famiglie.

**(ore 16,20)** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente. L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione del disegno di legge sulla proroga del termine per l'esercizio delle deleghe in materia di spettacolo. I relativi emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 10 di domani. La seduta sarà poi sospesa per riprendere alle ore 17 con la discussione del decreto-legge sulle liste d'attesa. Il termine per gli emendamenti è fissato un'ora dopo la trasmissione ai Gruppi del testo redatto dalla Commissione. L'esame del provvedimento continuerà nella giornata di giovedì 18, a partire dalle ore 9,30 e fino alla sua conclusione. Il previsto *question-time* di giovedì 18 non avrà luogo. Nelle settimane successive, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno discussi i seguenti decreti-legge: la prossima settimana, a partire dalle ore 11 di martedì 23 e fino a venerdì 26 luglio, se necessario: sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico; semplificazione edilizia e urbanistica; ricostruzione e protezione civile. Nella settimana da lunedì 29 luglio fino a sabato 3 agosto, se necessario: materia penitenziaria e giustizia civile e penale. Sarà inoltre discusso il disegno di legge per la proroga del termine di adozione di testi unici in materia tributaria, ove approvato dalla Camera dei deputati. Nella settimana da lunedì 5 fino a venerdì 9 agosto, se necessario: infrastrutture e investimenti strategici; processo penale e sport; materie prime critiche di interesse strategico. Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis,* del Regolamento, sui disegni di legge sulla semplificazione e digitalizzazione di attività economiche

Presidente, io prendo la parola per fare, per suo tramite, un ennesimo appello al nostro Esecutivo affinché sia subito cancellata una decisione che disonora il Governo stesso, il nostro Paese e offende la storia d'Italia. La decisione a cui mi riferisco - abbiamo avuto già modo di parlarne un'altra volta in questo consesso, in occasione della presentazione di una nostra interrogazione di una nostra interrogazione - è quella relativa all'emissione, negli stessi giorni in cui è stato dedicato un francobollo all'onorevole Giacomo Matteotti, di un francobollo dedicato ad Italo Foschi, Italo Foschi, che è stato uno squadrista tra i più pericolosi nell'ambito del fascismo romano, protagonista

dell'omicidio di Giacomo Matteotti; fu, nel secondo processo sull'omicidio di Giacomo Matteotti, coimputato per fatti che vennero attribuiti all'organizzazione clandestina, la cosiddetta Ceka, responsabile di crimini efferati. E vorrei dire soprattutto - lo sottolineo con grande forza - che Italo Foschi, durante il periodo buio della Repubblica sociale italiana nel Nord Italia, collaborò attivamente con i nazisti nelle attività di persecuzione degli ebrei italiani, che vennero deportati nei campi di sterminio e che fecero la fine che purtroppo tutti conosciamo. Nonostante da molte settimane abbiamo segnalato quanto sia scandaloso questo tipo di decisione e nonostante abbiamo pensato, in un primo momento, si potesse trattare di una svista facile da rimediare, ordinando la distruzione del francobollo, tutto questo non è avvenuto: i francobolli continuano a circolare, continuano ad essere spedite lettere in questo Paese con affrancature dedicate a un criminale di siffatta portata. Penso che questo sia motivo di vergogna per tutta l'Italia. Ma c'è di più: la Consulta filatelica, che è l'organismo che comprende esperti della materia filatelica e che dà pareri sulle emissioni di francobolli, si è riunita il 20 giugno e all'unanimità ha dato un parere assolutamente contrario alla emissione di questo francobollo e favorevole al suo ritiro e alla sua distruzione. A quella riunione era presente la sottosegretaria Bergamotto, giorni dopo quella riunione - e questo rende la vergogna enorme - né la sottosegretaria Bergamotto, né il ministro Urso hanno ritenuto di dover dar corso a quel parere della Consulta filatelica reso all'unanimità. Oggi chiediamo, allora, con più forza di quella che abbiamo messo nelle richieste precedenti, che questa decisione che disonora il nostro Paese venga cancellata, che il Ministro prenda immediatamente l'iniziativa di ritirare il francobollo e lo faccia distruggere. Oppure, se non fa questo, che il Ministro o la sua Sottosegretaria abbiano perlomeno il coraggio di venire in quest'Aula a spiegarci come mai un persecutore di ebrei, uno squadrista violentissimo e un esaltatore dell'omicidio di Matteotti sia degno di essere l'intitolatario e il dedicatario di un francobollo emesso negli stessi giorni in cui ne è stato emesso uno

Signor Presidente, sono qui in quest'Aula per parlare nuovamente - come è capitato anche ad altri colleghi - della situazione nelle nostre carceri. notizia di oggi che qualche giorno fa si è spento all'ospedale Parini di Aosta un detenuto di soli quarantadue anni, che si era sentito male all'interno della casa circondariale di Brissogne nei pressi di Aosta, un detenuto che versava già da qualche tempo in situazioni di salute critiche. Questo accende ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, un faro sulla situazione dei nostri istituti di pena, che ormai sta diventando insostenibile. La scorsa settimana ci sono state oltretutto rivolte in diverse carceri, tra cui quelle di Aosta

tra gli agenti di Polizia penitenziaria. È, quindi, un allarme che dovrebbe davvero far venire i brividi a tutti noi; a noi che pensiamo che - come recita la nostra Costituzione - la pena debba avere un carattere riabilitativo e non punitivo. Invece, soprattutto negli ultimi tempi, anche

l'assistenza sanitaria ai detenuti, i quali soffrono per le carenze di spazio. Insomma, guardiamo un po' più in là del nostro naso. E, soprattutto, invito il Governo e la maggioranza ad avere un po' più a cuore gli aspetti

Signor Presidente, lo scorso 12 luglio è scomparso a Trento Alberto Ferrandi, nato a Rovereto nel 1941 e deputato del Partito Comunista Italiano nella IX e nella X legislatura. figlio di Giuseppe Ferrandi, avvocato socialista e divenuto parlamentare della I legislatura repubblicana, dopo aver partecipato alla Resistenza e al Comitato di liberazione nazionale. Alberto ereditò dal padre gli ideali dell'antifascismo e della lotta partigiana, nonché la consapevolezza della specificità del Trentino e dell'Alto Adige. Giovanissimo dirigente della Federazione giovanile socialista, passa poi al Partito Comunista Italiano, di cui diventa funzionario negli anni Sessanta. Nel 1975 viene eletto segretario della Federazione provinciale di Trento e successivamente assume l'incarico di segretario regionale fino alle elezioni in Parlamento. Il suo impegno politico e la sua concezione della politica e del ruolo dei partiti solo direttamente collegati al pensiero e all'azione di Enrico Berlinguer, in particolare nel tentativo di costruire, anche a livello locale, un compromesso storico che nascesse dal basso, nel dialogo tra le culture politiche della sinistra e del mondo cattolico. Queste aperture portarono il Partito Comunista del Trentino, e in generale la sinistra, a uscire da una condizione di minorità, provando così ad incidere sulla trasformazione delle istituzioni autonomistiche della società e del territorio.

Alla Camera dei deputati lo fece in particolare grazie al rapporto con Renato Zangheri, Capogruppo del Partito Comunista Italiano, e di Giorgio Napolitano. Ferrandi seguì le questioni dell'autonomia speciale e della sua attuazione fino al momento della quietanza liberatoria rilasciata dall'Austria. Ferrandi apparteneva a una generazione e a un mondo nel quale il primato della politica chiamava tutti i suoi attori a una abnegazione quasi assoluta; a un impegno che si inverava attraverso un confronto che sapeva essere aspro, ma mai irrispettoso; a una capacità di ascolto e di radicamento sociale coltivata giorno dopo giorno, a una costante ricerca intellettuale e alla legittima convinzione che la politica fosse una delle branche più nobili della cultura del sapere, di cui è stato uno degli interpreti più bravi. Per questo, oggi lo salutiamo certi che il suo esempio e il suo impegno rimarranno per sempre nella storia di questo Parlamento e del nostro territorio, dove c'è ancora tanto da lavorare per superare l'indifferenza verso la politica e, molto spesso, il disprezzo verso i politici.